vorrei specificare in premessa che la SudGest Aid, come correttamente evidenziato nell'atto, è una società consortile senza scopo di lucro di cui - lo specifico - non sono mai stata presidente e nella quale non ho mai avuto potere di firma dei contratti,

Sottolineo altresì che, allo stato attuale, mi trovo in aspettativa per incarico istituzionale. Per ciò che attiene invece ai pregressi legami con la società in discussione, relativi alle specifiche circostanze richiamate dall'interrogante,

Progetto per il reintegro di ex combattenti come agenti di sicurezza per le aree archeologiche di Cirene, Sabratha e Leptis Magna». Ai fini della realizzazione del progetto, era necessario svolgere uno studio sull'area per comprendere quale tipo di approccio si dovesse assumere in quella regione e in quel peculiare contesto ambientale. Lo studio quindi era finalizzato a individuare il posto migliore dove svolgere il progetto coinvolta era una società di sicurezza, con il compito di svolgere appunto le attività di valutazione sulla sicurezza del luogo ove andava realizzato il progetto. Nel merito del quesito, pertanto, alla luce dei succitati elementi d'informazione, mi auguro di aver soddisfatto l'esigenza informativa manifestata dai senatori interroganti, in merito alla necessità di chiarire con la massima sollecitudine i reali rapporti con la citata società consortile SudGest Aid. Grazie e viva l'Italia.

di dire che se è così preoccupata delle *fake news* che circolano sul suo ruolo e sul pregresso delle sue attività, non avrebbe dovuto attendere quattro mesi per dare "sollecita" risposta

è necessario innanzitutto premettere che l'agglomerato di Pescasseroli è oggetto della procedura d'infrazione 2009/2034, avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano. La motivazione che ha determinato l'avvio nel 2009 della citata procedura è «l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 (sistemi fognari), 4 (sistemi di trattamento), 5 (sistemi di trattamento più spinti) e 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE». In particolare, l'agglomerato di Pescasseroli risulta essere in violazione degli articoli 4, 5 e 10 della direttiva. In considerazione della necessità di giungere, nel più breve tempo possibile, alla risoluzione del contenzioso comunitario e per dare impulso alla realizzazione degli interventi negli agglomerati coinvolti, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proceduto, nel 2015, alla nomina di commissari straordinari, successivamente sostituiti da un unico commissario straordinario di Governo. Per quanto concerne, nello specifico, la realizzazione dell'impianto in questione, secondo quanto riferito dalla Regione Abruzzo, dall'ente parco e dal predetto commissario straordinario unico, l'intervento «Disinquinamento del Lago di Barrea: sistema depurativo a servizio dei Comuni di Pescasseroli e Opi, delocalizzato in località "Peschiera" - I stralcio; Intervento relativo al depuratore consortile e al collettamento dei reflui del Comune di Pescasseroli» è articolato in tre stralci funzionali, per complessivi 6,75 milioni di euro. Il Comune di Pescasseroli, con delibera del 15 novembre 2011, ha approvato il progetto preliminare del primo stralcio che prevedeva l'ubicazione dell'impianto di depurazione nella località Colle della Regina. Successivamente, con delibera del 5 giugno 2014, il Comune ha proposto la riallocazione dell'impianto di depurazione dalla località Colle della Regina all'area in località Peschiera. La riallocazione si riteneva opportuna in quanto la sede originariamente scelta risultava essere troppo interna alla piana, rendendo necessaria la realizzazione di un collegamento viario, ed eccessivamente vicina al fiume Sangro. Ciò avrebbe comportato problematiche di sicurezza connesse ai periodi di piena e di secca del predetto fiume. In data 11 settembre 2014, il progetto definitivo di primo stralcio è stato sottoposto al Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale Il 17 febbraio 2015, il Presidente del Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise ha inviato una nota al Comitato, con cui esprimeva parere negativo all'approvazione della VIA. Conseguentemente, nel marzo 2015 il CCR-VIA ha espresso giudizio di preavviso negativo. Nello stesso mese di marzo 2015 si è tenuto, presso il Consiglio regionale, un incontro per discutere la questione relativa alla localizzazione dell'impianto di depurazione. I presenti alla riunione, preso atto del preavviso di rigetto espresso dal CCR-VIA, concordavano di approvare, quale ubicazione alternativa del depuratore, la proposta espressa dal Consiglio comunale di Pescasseroli relativamente alla località Peschiera. Il 25 marzo 2015 si è tenuta apposita riunione presso il Ministero dell'ambiente, nel corso della quale l'Ente parco ha ribadito il proprio orientamento di riallocare l'impianto di depurazione dalla località Colle della Regina alla località Peschiera. A seguito del preavviso di rigetto espresso dal Comitato in merito all'ubicazione originaria, l'ATI aggiudicataria ha, quindi, predisposto il progetto esecutivo di perizia del primo stralcio conseguente al cambiamento di ubicazione. Il progetto mantiene immutato il quadro economico di 4.150.000 euro e pertanto l'intervento non presenta criticità finanziaria. Nel 2017 il progetto è stato sottoposto al commissario straordinario unico che, il 7 settembre, ha stipulato una specifica intesa con la Regione Abruzzo, l'Ente d'ambito e il soggetto attuatore. A ciò si aggiunga che, tra le prescrizioni poste per la realizzazione dell'opera, è stato previsto un sistema di alimentazione supplementare delle pompe per ovviare ad eventuali malfunzionamenti. La SACA SpA, soggetto gestore del servizio idrico integrato, e stazione appaltante dell'intervento di realizzazione dell'impianto depurativo a servizio dell'agglomerato di Pescasseroli, ha ridefinito il cronoprogramma dei lavori, prevedendo data di inizio lavori il 2 ottobre 2017 e come data di ultimazione lavori il 17 marzo 2019; come data di entrata in funzione per raggiunta conformità il 2 novembre 2019. Alla luce delle informazioni esposte, risulta dunque che l'intervento di cui trattasi è in avanzato stato di realizzazione e che l'*iter* procedurale seguito, pur nell'urgenza che la situazione impone in seguito al commissariamento, ha tenuto in considerazione le esigenze delle diverse realtà territoriali coinvolte. Ad ogni modo, si rassicura che il Ministero dell'ambiente continuerà a svolgere la propria attività di monitoraggio e manterrà alto il livello di attenzione sulla questione.

salita, con tutto quello che ciò comporta per quanto riguarda l'aggravio non solo dei costi, ma anche il problema delle pompe di sollevamento. Vorrei far presente che, che, come già anche nella risposta in qualche modo si prevede, in caso di malfunzionamento delle pompe di sollevamento il risultato sarebbe che tutte le acque nere del comune di

Vanno benissimo la sorveglianza e il controllo da parte del Ministero dell'ambiente ma purtroppo questi problemi tecnici, che potrebbero avere un impatto ambientale devastante per

passa anche parallelamente alla piana alluvionale del fiume, con tutto quello che ciò comporta, variando spesso anche il suo percorso. Considero quindi la risposta non sufficiente e non soddisfacente per quanto ci riguarda e comincio ad allarmarmi seriamente rispetto a quelli che potrebbero essere i risultati finali. Per rispondere ad una procedura di infrazione, anche giusta, bisognava però mettere in atto delle scelte anche dal punto di vista tecnico e di collocazione

Signor Presidente, con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta che, per quanto concerne l'incendio verificatosi lo scorso giugno presso la Nappi Sud di Battipaglia, sebbene dai primi rilievi si sia accertato che il rogo non ha interessato i rifiuti ma il capannone industriale con i macchinari ed alcuni materiali legnosi, il Comune di Battipaglia, a fini esclusivamente cautelativi, ha emanato, nell'immediatezza dell'evento, un'ordinanza urgente disponendo, per tutti i residenti, l'allontanamento dalle case e dagli edifici ricadenti entro un raggio di 100 metri fino al termine delle operazioni di spegnimento. protezione ambientale (ARPAC), le squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Più in particolare, secondo quanto riferito dall'ARPAC, dall'esito analitico del campionamento di terreno *top soil* *top soil* per la verifica suolo è emerso che i campioni di terreno C1 e C3 presentavano valori di concentrazione inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione per i siti ad uso commerciale e industriale e il campione C2 di terreno presentava valori di concentrazione inferiori alle soglie di contaminazione per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Anche per quanto attiene la ricerca dei parametri PCB,

In riferimento ai superamenti per il parametro berillio nei campioni di suolo denominati C1 e C3, l'ARPAC ha ritenuto che gli stessi possano essere attribuiti a valori di fondo naturale. Inoltre, dalle risultanze analitiche dei campionamenti utili alla ricerca nell'aria di idrocarburi policiclici aromatici effettuati tra il 25 e il 26 giugno, ARPAC non ha evidenziato criticità in merito all'andamento della qualità dell'aria. In merito agli aspetti prettamente sanitari inerenti agli incendi in questione, la ASL competente ha riferito che non sono pervenute segnalazioni di fastidi o disagi da parte della popolazione circostante. La ASL ha inoltre attivato uno specifico monitoraggio sulla produzione agricola e sugli allevamenti. Per quanto attiene, più in generale, il verificarsi nella Regione Campania di episodi incendiari, il Ministero dell'interno ha segnalato, da parte sua, di aver adottato apposita circolare del 13 luglio 2018 in seguito alla quale è stato deciso di sottoporre i siti regionali ad una più assidua attività di controllo e di inserirli, quali obiettivi da vigilare, nell'ambito dei piani di controllo

nonché al sindaco di Salerno, alla più ampia collaborazione per il soddisfacimento delle richiamate esigenze. I predetti enti hanno assicurato la loro tempestiva attivazione presso le società partecipate che gestiscono i siti di stoccaggio per l'adozione delle l'adozione delle necessarie misure di difesa passiva nelle strutture interessate. Ferme restando le considerazioni esposte si segnala che, considerata la frequenza degli episodi di combustione, nel mese di marzo scorso il Ministero dell'ambiente ha provveduto a pubblicare una circolare recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi», con l'obiettivo di prevenire l'innesco d'incendi e favorire la corretta gestione degli stoccaggi presso gli impianti di trattamento dei rifiuti. Il Ministero ha avviato, inoltre, congiuntamente al comando dei Vigili del fuoco e alle autorità regionali, le attività finalizzate all'aggiornamento delle linee guida per una gestione in sicurezza dei rifiuti. La Regione Campania, a sua volta, ha fatto presente di aver avviato, con delibera n. 705 dell'ottobre scorso, un rafforzamento delle attività di pattugliamento per i siti ritenuti maggiormente sensibili e vulnerabili e di aver previsto, con legge regionale n. 29 del 2018, l'elaborazione di linee guida volte all'implementazione di misure di prevenzione antincendio

di un piano di emergenza interna al fine, tra l'altro, di controllare e circoscrivere gli incidenti e provvedere al ripristino dell'ambiente; la norma prevede altresì che, al fine di limitare gli effetti dannosi di incidenti rilevanti, il prefetto predispone un piano di emergenza esterna e ne coordina l'attuazione. Inoltre, nel recente protocollo d'intesa sul Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti sono state introdotte, tra l'altro, specifiche misure volte ad intensificare il coordinamento delle attività di prevenzione, gestione dell'evento e ripristino delle aree coinvolte dagli incendi, allo scopo di aumentare la sicurezza del territorio e garantire la tutela dell'ambiente

signor Sottosegretario, devo necessariamente dichiararmi insoddisfatto della risposta. Questo non per la sua cortesia, ma perché, per quanto viene riferito dalle relazioni, mi risulta assolutamente incredibile che gli eventi che si sono verificati a Battipaglia, che è la seconda città della Provincia di Salerno, in occasione del mese di giugno non abbiano destato allarme sociale e che i dati possano presentare una situazione di sicurezza per quello che è avvenuto, che è stato un incendio veramente spaventoso presso la Nappi Sud, così come grande preoccupazione ha destato l'incendio che si è verificato presso lo Stir di Battipaglia. una città che è stata martoriata da scelte politiche che ne hanno fatto realmente l'immondezzaio della Provincia di Salerno. Sono all'ordine del giorno i disagi che vivono i cittadini. Sono all'ordine del giorno le preoccupazioni che vengono portate avanti dai comitati cittadini e raccolte dall'amministrazione comunale. Mi sarei aspettato un maggior coraggio da parte del Governo nella risposta a quello che stiamo verificando in Campania è veramente paradossale. Il ciclo dei rifiuti in Campania non è assolutamente chiuso. La Campania vive un'emergenza, e Battipaglia è uno dei punti di maggiore criticità, per effetto delle scelte di cui La Regione Campania del governatore De Luca ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza ad affrontare e a risolvere il problema.

Già nel mese di marzo denunciavo che ci si avviava verso una nuova emergenza e i fatti, anche quelli degli ultimi giorni, dicono esattamente questo. Però mi sia consentito di dire che noi non possiamo tornare indietro di vent'anni in una discussione assolutamente ideologica (termovalorizzatore sì, termovalorizzatore no) quando abbiamo queste situazioni che non vengono minimamente affrontate. C'è un'altra situazione di gravissima emergenza a Torre del Greco con muri di immondizia alti tre metri e abbiamo assistito, nello scorso fine settimana, ad un teatrino interno alla maggioranza di Governo; abbiamo assistito ad una visita a Caserta che io non ho capito con quali decisioni si sia conclusa in termini operativi per affrontare l'emergenza e chiudere questo benedetto ciclo dei rifiuti in Campania. allora rivolgere un appello al Governo, signor Sottosegretario, attraverso la sua cortesia: in attesa della decrescita felice o infelice, in Campania continua a vigere la stabilità del provvisorio. È necessaria una iniziativa politica forte del Governo centrale che vada a risolvere il problema perché chi è stato e chi è causa del male e di questa situazione indecorosa certamente non può esserne la soluzione e parlo del governo regionale di De Luca e delle istituzioni locali.

senatore Misiani, nel rispondere alla sua interrogazione evidenzio preliminarmente quanto già rappresentato l'8 novembre presso la 7a Commissione in in risposta ad analogo quesito e cioè che l'amministrazione è in procinto di bandire, in quanto è imminente l'autorizzazione, la procedura concorsuale che permetterà di ovviare alle difficoltà gestionali verificatesi fino ad oggi a causa della carenza di organico nel profilo professionale dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, attraverso il loro reclutamento, come disposto dall'articolo 1, comma 605, della legge di bilancio per l'anno 2018. In base a quanto prescritto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, alla stessa procedura concorsuale potranno partecipare coloro che sono in possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche, sociali ed amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti. Segnalo altresì che saranno ammessi anche coloro che hanno svolto per tre anni di servizio negli ultimi otto le mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in assenza del titolo di studio richiesto. Con specifico riguardo alla deficienza di soluzioni alternative da lei richiamate, intendo rassicurarla sul fatto che nelle more dell'espletamento del concorso, per far fronte alla carenza di personale in servizio, la contrattazione collettiva prevede il ricorso ad una pluralità di istituti. Scendendo più nel dettaglio, innanzitutto, qualora a seguito delle procedure di utilizzazione dell'assegnazione provvisoria residuino posti vacanti e disponibili la sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) è effettuata in conformità con quanto disposto all'articolo 14 dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo del 2018 per l'anno scolastico 2018-2019. In tal caso l'incarico è prioritariamente assegnato all'assistente amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola, titolare della seconda posizione economica. Qualora, invece, vi siano più assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica disponibile a sostituire il DSGA, il dirigente scolastico emana un bando interno di selezione per l'individuazione dell'assistente amministrativo cui conferire l'incarico. Inoltre, se nell'istituzione scolastica non vi sono assistenti amministrativi con la seconda posizione economica, la sostituzione del DSGA può essere affidata all'assistente amministrativo titolare della prima posizione economica o di incarico specifico; questi ultimi, però, diversamente da quelli con la seconda posizione economica, non sono obbligati alla sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico nella scuola di servizio. Da ultimo, nel caso di mancata sostituzione del DSGA con un soggetto interno all'istituzione scolastica l'Ufficio scolastico regionale predispone un elenco di assistenti amministrativi che abbiano manifestato la propria disponibilità ad accettare un incarico a tempo determinato nel profilo professionale DSGA. Queste procedure di interpello hanno prioritariamente valenza provinciale ma possono assumere anche carattere regionale o, in ultima analisi, nazionale. Per concludere, aggiungo che, nell'eventualità in cui anche l'interpello fuori Regione

Signor Presidente, c'era un buon adagio nella pubblica amministrazione (me l'ha insegnato un mio vecchio maestro): mai mettere un architetto a fare l'assessore all'urbanistica.

Quando ho scorto le nomine di questo Governo e ho trovato troppi tecnici al posto di politici, mi sono abbastanza preoccupato. La mia preoccupazione si è resa palpabile in varie occasioni, non ultima questa mattina, perché ci si limita all'analisi delle questioni dal punto di vista tecnico, discendendo sempre da pareri altrettanto tecnici, che provengono dall'interno dei Ministeri. Ora, non vorrei far aleggiare in quest'Aula il fantasma di Rocco Casalino, che protestava contro i tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze

che sono dietro gli alunni. Caro professore, dietro agli alunni ci sono le famiglie, che ogni mattina in 2.400 scuole italiane - anche stamani - trovano

ha sanato questa situazione e ha «patteggiato» in una logica di scontro amministrativo-giurisdizionale la posizione delle DSGA, assumendo nel ruolo superiore anche coloro i quali non avevano il titolo

quando è entrato al Ministero probabilmente ha azzerato la memoria. Vi do un consiglio: andate sul territorio, parlate con chi usufruisce dei servizi e tenete in considerazione queste persone che per anni hanno sopperito ad una mancanza istituzionale dello Stato, che li ha lasciati in trincea senza neppure ringraziarli. Signor Presidente, parliamo di una situazione molto difficile, ma ampiamente prevedibile, che ha riguardato, ad inizio anno scolastico, 485 scuole in Lombardia, moltissime in tutta Italia, e 79 su 139 in Provincia di Bergamo. Senza il DSGA c'è la paralisi contabile e amministrativa delle scuole, che non possono pagare i supplenti e i fornitori, non possono stipulare l'assicurazione per i dipendenti, non possono gestire i piani per il diritto allo studio e i progetti. Ripeto, la paralisi totale. Noi prendiamo atto della risposta del Sottosegretario circa l'imminente indizione di un concorso. Sono passati undici mesi dall'approvazione della legge di bilancio 2018; undici dalla norma che ha autorizzato l'avvio di questo concorso. Speriamo che sia arrivato il tempo. Il punto è: cosa facciamo oggi? In Provincia di Bergamo ci sono ancora quattro scuole prive di DSGA. Sono andate a vuoto le sollecitazioni nei confronti degli assistenti amministrativi; alcuni è da più di dieci anni che si fanno carico di questa funzione senza riconoscimenti economici, assumendosi responsabilità non loro. Gli interpelli sono andati a vuoto. Ne è stato fatto un ultimo in Provincia di Bergamo per tutta Italia; scade il 24 novembre ma, sentendo oggi la responsabile dell'ufficio scolastico provinciale, non c'è motivo per essere ottimisti. Io chiedo a lei, signor Sottosegretario, se non sia il caso di introdurre una norma per autorizzare una reggenza da parte dei DSGA, analogamente a quanto previsto con i dirigenti scolastici, cioè prevedere un ulteriore strumento che permetta di risolvere subito, nelle more dell'indizione del concorso, una situazione che è francamente insostenibile e che indebolisce un servizio pubblico essenziale per le famiglie e gli studenti.

hanno la funzione dei vecchi applicati di segreteria, degli assistenti amministrativi, lei si dovrebbe chiedere perché in questo momento vi è una risposta negativa.

modo si creerebbe un'aspettativa e si darebbe un riconoscimento a coloro che per anni si sono assunti oneri e responsabilità senza avere assolutamente nulla in cambio, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista della progressione di carriera. Mi auguro, quindi,

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderà il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali,

hanno espresso forte contrarietà allo schema di decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto ridurrebbe sensibilmente gli incentivi per gli impianti con una potenza inferiore a un megawatt. In particolare, però, si lamenta l'esclusione quasi totale dagli incentivi del settore idroelettrico: in questo modo verrebbe meno uno strumento di sostegno all'economia piccola, all'economia circolare e all'economia montana, un abbassamento delle difese idrogeologiche legate alla regolazione dei flussi e delle opere di compensazione ambientale. Inoltre, la mancata possibilità e convenienza ad accedere a una tariffa incentivante adeguata potrebbe comportare una drastica riduzione di entrate autonome per le comunità locali, con evidenti implicazioni per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Noi crediamo invece che la strategia energetica nazionale non possa fare a meno di questo settore che contribuisce all'economia nazionale in termini energetici, ambientali, economici e sociali. Per questo si chiede al signor Ministro di sapere se non ritenga opportuno riconsiderare i criteri e i contingenti di potenza messi a disposizione per gli impianti idroelettrici e, più in particolare, se non ritenga necessario favorire l'accesso agli incentivi degli impianti idroelettrici già esistenti e validamente iscritti in posizione non utile nel Registro 2016, eventualmente prevedendo l'accesso diretto alla tariffa incentivante o a eventuali premi. se non ritenga di garantire, a favore delle piccole e medie centrali idroelettriche, l'accesso diretto agli incentivi per nuove costruzioni, ampliamenti e interventi di ristrutturazione con procedure semplificate. se non ritenga di incentivare anche i nuovi impianti su corsi d'acqua a tratti liberi, considerando che nel procedimento di rilascio della concessione idroelettrica viene valutato e garantito che l'impianto idroelettrico progettato non abbia effetti negativi sulla buona qualità del corso d'acqua.

da procedure di ammissione e di riconoscimento che garantiscono un meccanismo di controllo della spesa, sia in termini di tetto complessivo da non superare, sia in termini di allocazioni annue a ciascuna tecnologia. La bozza di provvedimento trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico l'8 novembre 2018 alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere di competenza mira a dare continuità all'installazione di nuova capacità rinnovabile, anche in considerazione dell'ambiziosa bozza di Piano energia e clima che stiamo redigendo, con il quale puntiamo a conseguire un raddoppio in poco più di dieci anni della produzione di energia rinnovabile. In questo contesto, in mancanza di un controllo della spesa per incentivi si rischierebbe di gravare troppo sulle bollette energetiche delle famiglie e delle imprese. Per questo abbiamo scelto - ciò vale per tutte le tecnologie e le dimensioni di impianto - di non prevedere più l'accesso diretto agli incentivi, ma di riconoscere l'incentivo solo ai progetti selezionati a seguito di procedure di asta o registro, attraverso l'utilizzo di criteri competitivi o requisiti di priorità. In questo modo, infatti, in caso di eccesso di domande, possono essere individuati gli impianti più meritevoli da un punto di vista ambientale o dell'efficienza (intesa quale rapporto tra spesa per incentivi ed energia pulita prodotta). È noto che, con specifico riferimento alla tecnologia idroelettrica, la bozza di decreto ammette ad incentivazione solo quegli impianti che non effettuano prelievi aggiuntivi dai corpi idrici oggetto di derivazione,

questo - di particolare vulnerabilità, che vede l'Italia soggetta a diverse procedure di infrazione da parte della Commissione europea per la violazione della direttiva 2000/60/CE La tutela dell'ambiente è per noi un valore irrinunciabile. Bisogna anche ricordare le numerose proteste pervenute nell'ultimo anno da parte di vari territori intensamente interessati dalla nascita di piccoli impianti idroelettrici, che hanno lamentato la mancanza di una programmazione nell'uso delle risorse, fattore che, insieme all'elevato livello degli incentivi e al meccanismo dell'accesso diretto, ha finito per rendere troppo forte la pressione sull'ambiente. Abbiamo il dovere di tenere in fortissima considerazione la voce dei territori. La previsione contenuta nello schema di decreto non consente di ammettere agli incentivi i progetti inclusi nel Registro 2016 in posizione non utile, dal momento che per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per tali casi non sono state applicate le linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche e le linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale. Il tema sarà comunque discusso con le Regioni e gli enti locali nel passaggio del testo in Conferenza unificata.*(Applausi dal

cereali canadesi contaminati da atrazina, che è tra le 99 sostanze chimiche vietate in Italia e perfettamente legali in Canada (che, peraltro, aspetti più pericolosi di quel Trattato). Sa anche perfettamente, Ministro, che il nuovo trattato di liberalizzazione commerciale, sottoscritto da Canada, Stati Uniti e Messico, il nuovo NAFTA, ha cambiato molte regole del mercato interno canadese, a partire dall'origine delle merci; per cui non sarà più possibile individuare

lei sa, è stato costituito un intergruppo parlamentare, già dalla scorsa legislatura e riconfermato anche in questa, formato da parlamentari di tutti i Gruppi che si oppongono alla ratifica del CETA. Voglio sapere da lei, Ministro e Vice *Premier*,

La *task force* del libero scambio, istituita presso il MISE nello scorso agosto, è un meccanismo di lavoro aperto al contributo di tutte le parti sociali, volto a valutare, su base analitica e non pregiudiziale, l'impatto dei trattati di libero scambio in fase di negoziazione o di ratifica da parte dell'Unione europea. Resta nostro obiettivo dimostrare tutti i motivi per cui questo Trattato, così come ci è stato proposto, non sia ratificabile. Abbiamo il dovere di tutelare innanzi tutto gli agricoltori italiani, gli imprenditori che operano nella filiera agroalimentare, la cui attività deve essere protetta, e i diritti dei consumatori italiani. Gli studi del gruppo operativo saranno mirati a focalizzare sia i benefici che i picchi negativi degli accordi, essenzialmente a protezione delle fasce sociali più deboli, colpite dal processo di globalizzazione, permettendo in tal modo al Governo di identificare il migliore approccio per rendere l'Italia più competitiva nel contesto internazionale, garantendo allo stesso tempo maggiore equità e giustizia sociale. La *task force* che si è riunita per la terza volta, come noto, martedì scorso al MISE, è stata incentrata sul trattato CETA. Il dibattito si è focalizzato sulla tematica delle indicazioni geografiche, analizzando la tutela prevista nell'accordo, con lo scopo metodologico di avere sessioni speciali sul CETA, ognuna dedicata a un tema specifico del trattato. In questa sede si è ritenuto di estendere la discussione in merito alla nuova normativa interna canadese in materia di indicazioni geografiche, che adotta i principi del CETA modificando il Trademark act canadese e che - consentendo di registrare con facilità nuove indicazioni non comprese già tra quelle protette dal Trattato - può offrire un ulteriore grado di tutela alle nostre indicazioni geografiche, nonché sulla possibilità esistente di presentare reclami contro le usurpazioni e le contraffazioni nel mercato canadese (sia di provenienza canadese che estera). Nelle prossime settimane, si terranno ulteriori sessioni su questo Trattato e successivamente sui trattati di libero scambio attualmente in fase di negoziazione anche avanzata da parte dell'Unione europea. In attesa dei risultati dei lavori della *task force,* il Governo, così come previsto nel contratto, si opporrà agli aspetti che comporteranno un eccessivo affievolimento della tutela dei diritti dei cittadini, oltre a una lesione della corretta e sostenibile concorrenza sul mercato interno.

*(FdI)*. Signor Ministro, sono noti i disagi provocati ai cittadini a causa della riforma dei tribunali, che ha chiuso circa mille uffici, al fine - dichiarato - di rendere i tribunali più efficienti e meno costosi. In particolare, la riduzione dei tribunali non ha tenuto in considerazione alcune specificità territoriali, quali la conformazione orografica e la situazione dei collegamenti infrastrutturali, il tasso di litigiosità, quello di criminosità e la presenza di istituti penitenziari nei pressi dei tribunali, alcuni dei quali persino in ampliamento. Nel contratto di Governo si legge che occorre modificare la riforma del 2012, con l'obiettivo di riportare tribunali, procure e uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese. poche righe, che tuttavia sembrano legittimare l'aspettativa che il Governo voglia ripristinare i cosiddetti tribunali minori, dando seguito a una delle tante promesse elettorali. Nonostante tale impegno scritto, nulla è stato fatto finora. Al contrario, le dichiarazioni rese dal ministro Bonafede a Catania il 5 ottobre e alla Camera il 31 dello stesso mese mostrano l'intenzione di non riaprire i tribunali soppressi, ma di surrogarli con uffici di prossimità che non servono a niente, come ha dimostrato anche la fallimentare sperimentazione di Tolmezzo. Tali dichiarazioni hanno peraltro provocato una reazione uguale e contraria del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che ha richiamato l'alleato di Governo al rispetto dei patti sulla materia. Come ha evidenziato la Commissione europea per l'efficienza della giustizia, nelle condizioni di accesso a un sistema giudiziario di qualità, dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana o per una che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresenta una situazione problematica, che può influire sul diritto di equo accesso alla giustizia. Tale diritto viene di fatto negato quando, per effetto delle soppressioni, le distanze dai Comuni più lontani verso la sede accorpata arrivano addirittura ai 112 chilometri di Sulmona, ai 90 di Mistretta, ai 77 di Vasto, e così via, con tempi di percorrenza fino a 80, 90, 115 minuti. stata fortemente sottovalutata la componente orografica dei territori interessati: solo per citare le altitudini medie più elevate, Nicosia arriva a 788 metri su livello del mare, Sulmona a 780, Avezzano 778 e Ariano Irpino a 617. Il Ministro non ha dato alcuna risposta alla richiesta di soluzioni alternative presentate da Regioni ed enti locali, come ad esempio quelle per salvaguardare i tribunali abruzzesi, che sono tuttora aperti fino al 2020, solo grazie a una deroga a causa dei terremoti che si sono succeduti. Si tratta di una situazione tragica e al limite del grottesco. Che Stato miserabile è quello nel quale i cittadini devono augurarsi un terremoto o una calamità naturale per vedersi riconosciuta l'utilità della presenza di tribunali, ospedali, caserme e uffici pubblici?

Oltretutto ora c'è la commissione Rordorf che ha preparato una bozza per la riforma dei tribunali concorsuali che interverrà ulteriormente. Domandiamo quindi al Governo quali sono le sue intenzioni riguardo alla soppressione dei tribunali; come intende garantire il diritto di equo accesso alla giustizia di ogni cittadino; se vuole sottoscrivere le convenzioni con le Regioni e gli enti locali e quando riceverà il coordinamento dei tribunali soppressi costituitosi a luglio scorso.

rispondo sulla base delle indicazioni che mi sono state fornite dal Ministero della giustizia. La distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale non può prescindere dalle peculiarità delle singole aree geografiche che lo compongono sia in relazione alla qualità e alla quantità del contenzioso e della densità criminale che sul piano della dislocazione logistica, anche tenuto conto del non secondario aspetto delle distanze chilometriche, dei collegamenti e delle infrastrutture. Uno sforzo di razionalizzazione deve essere teso anche a favorire logiche di specializzazione del personale di magistratura che rischiano di essere frustrate da un'eccessiva frammentazione degli uffici giudiziari. Devo rassicurare gli onorevoli interroganti sul fatto che l'azione di questo Governo è assolutamente ispirata ai canoni della prossimità territoriale. Ne è esempio concreto la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del termine di temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia, Portoferraio e Lipari, sede quest'ultima inclusa nel territorio siciliano a cui l'interrogante fa espresso riferimento. Quanto alle sedi giudiziarie abruzzesi oggetto di soppressione, il regime di proroga fino al 2020 offre, ad oggi, una utile parentesi temporale in cui sviluppare ogni riflessione sulle possibili soluzioni da adottare in futuro, sempre nell'ottica della sensibilità alla prossimità territoriale. Con lo schema di decreto legislativo recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", inoltre, si è operata la precisa scelta di mantenere in vita tutte le attuali sezioni specializzate, escludendo qualsiasi ipotesi di soppressione. Devo però aggiungere che occorre un ripensamento concettuale della geografia giudiziaria in forza del quale prendere atto che l'esercizio della giurisdizione è solo un segmento del più vasto complesso sistema giustizia, che passa anche attraverso una serie di adempimenti e servizi. È proprio in questo solco che si muove il progetto degli uffici di prossimità, elaborato nell'ottica di potenziare l'equo accesso alla giustizia mediante la costituzione di una rete integrata di servizi al cittadino, concepita quale strumento di raccordo non solo per gli uffici giudiziari, ma anche con ogni altra struttura istituzionale con cui l'utente deve interfacciarsi per poter tutelare in sede giudiziaria i propri interessi. Si tratta di un progetto che prevede la dislocazione su tutto il territorio nazionale di veri e propri sportelli dedicati al cittadino, affatto surrogatori dei tribunali, offrendo rispetto ad essi servizi diversi e ulteriori, quali l'invio di dati telematici, il ritiro di notificazioni e comunicazioni, la ricezione di atti e documenti, senza dover affrontare alcuno spostamento logistico. Il progetto, del resto, verrà presentato alle Regioni, proprio qui in Senato, il prossimo 11 dicembre e sarà questa l'occasione per un confronto

sua risposta è assolutamente insoddisfacente e negativa. Ha usato giri di parole per non dichiarare la verità e cioè che non volete riaprire tali tribunali

la geografia per capirlo. Cito solo il caso dell'Abruzzo: basta osservare la linea di demarcazione tra i tribunali soppressi e quelli che rimangono in piedi per capire che mezza Regione rimane senza un solo tribunale, quando la Regione vicina, nello stesso territorio, ne ha almeno tre e la Provincia confinante di Frosinone altri due. Non capisco come si possa dire che in quel territorio ci sia un equo accesso alla giustizia, quando ci vogliono due ore dal Comune più remoto

a quello di Asti, che è in altra Provincia, ha contraddetto in quel momento la previsione legislativa secondo cui la ridefinizione dei circondari di tribunale doveva avvenire preferibilmente nell'ambito della stessa Provincia, tenuto conto anche del fatto che nella Provincia di Cuneo, terza per ampiezza territoriale in Italia, sono stati soppressi ben tre dei quattro tribunali esistenti e quello di Cuneo - unico rimasto al di là dell'efficienza del personale, ha un sovraccarico di lavoro che lo raccomando. La riforma della geografia giudiziaria ha previsto poi la soppressione del tribunale di Alba senza tenere alcun conto del fatto che in Piemonte, sotto la corte d'appello di Torino, che raccoglie due Regioni (Piemonte e Valle d'Aosta) erano 17 i tribunali presenti e quello di Alba rappresentava il quarto in graduatoria come volume di lavoro,

La popolazione della Provincia di Cuneo è di 592.000 abitanti e per avere due tribunali bisognava che la popolazione fosse di oltre 700.000 abitanti, che si potevano comprendere con la parte Sud di Torino, che era già parte integrante del tribunale di Alba. Ricordo anche il fatto che il tribunale di Alba ricopre una zona dove è presente anche la casa circondariale, con oltre 200 detenuti. Vogliamo pertanto chiedere al Ministro se non reputi doveroso adoperarsi per una riapertura di questo tribunale, al fine di garantire una migliore operatività e un miglior servizio della giustizia in questo territorio. Ricordo che in Provincia di Cuneo vi sono 690.000 abitanti, 80.000 imprese iscritte alla Camera di commercio, con un tasso di disoccupazione del 5 per cento, il che significa che c'è operatività e il territorio ha bisogno di risposte veloci anche dal punto di vista amministrativo. Poiché poi abbiamo diverse segnalazioni di tribunali che non verranno riaperti, chiedo quali sono i tempi

sul territorio in termini economici e logistici. In occasione di un recente convegno, il ministro Bonafede ha già avuto modo di raccogliere personalmente le istanze dei cittadini di Alba, proprio con riferimento alla chiusura del tribunale in questione. istanze debbono tuttavia necessariamente inserirsi da un lato nel quadro complessivo relativo alla Provincia di Cuneo, come sottolineato, dall'altro lato nelle risultanze organizzative dell'avvenuto accorpamento, che non fanno che non fanno rilevare criticità sotto questo aspetto. Il Ministero della giustizia ha inoltre chiesto al primo cittadino di Alba contezza del funzionamento dell'ufficio di prossimità già esistente sul territorio, tema sul quale si attende una relazione dettagliata per verificare le possibili e le ipotesi di un ulteriore intervento. Tanto premesso, il Ministero della giustizia raccoglie la sfida riguardante la verifica dell'efficienza della macchina giudiziaria, riservando una completa attenzione alle esigenze dei cittadini, del territorio ed alla necessità di voler garantire una razionale e capillare rete di strutture di riferimento a garanzia della legalità. L'impegno siglato nel contratto di Governo, con riguardo alla rivisitazione della riforma della geografia giudiziaria, si traduce, pertanto, nella necessità di verificare di volta in volta la razionalità delle scelte in precedenza operate circa la dislocazione dei tribunali e le opzioni di accorpamento realizzate. Proprio nella direzione di un simile impegno si potrà, in prima battuta, pensare ad un potenziamento dell'ufficio di prossimità esistente ad Alba, incrementandone i servizi in favore del bacino di utenza di riferimento, senza lasciare preclusa, ove possibile e necessaria, ogni ulteriore scelta organizzativa del caso. La particolare sensibilità con la quale si affronta il tema sottoposto dall'onorevole interrogante ha comunque portato il Governo a determinarsi, in taluni casi, verso soluzioni organizzative ritenute più efficaci a gestire le istanze di giustizia di determinati territori, come è accaduto con il cosiddetto milleproroghe 2018 e con lo schema di decreto legislativo recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza". La visione concreta ed operativa del sistema giustizia che si intende realizzare, persegue, infatti, l'obiettivo di accrescere il livello di servizi offerti in sede locale all'utenza con la messa a regime degli uffici di prossimità proprio per garantire un efficace presidio di giustizia sul territorio. Inoltre, si sta realizzando un'attività di coordinamento con i Comuni finalizzata a raccogliere informazioni presso gli uffici giudiziari interessati dai provvedimenti di riorganizzazione accorpanti e dei territori di beni e/o apparecchiature esistenti presso gli uffici soppressi. In ogni caso, concludendo, si sottolinea che ogni modifica organizzativa e di distribuzione degli uffici sul territorio non può prescindere dal bilanciamento tra i vari interessi coinvolti nell'ottica di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficacia della giustizia al servizio del cittadino,

Signor Ministro, grazie per la risposta. Comunque, noi abbiamo più volte lamentato, sia come ordini forensi del territorio sia come amministratori dei Comuni (le ricordo che è una realtà di 250 Comuni, molto dimensionata sul territorio), che tale territorio ha bisogno di una attività amministrativa importante. Mi piacerebbe molto che il signor Ministro valutasse con attenzione quanto accaduto dal 2011 ad oggi, rivedendo praticamente questa politica di decentramento, che è stata ridimensionata nel tempo, laddove la chiusura di questi tribunali ha creato dei problemi,

15,34)** (*Segue* BERGESIO). Occorre ribadire, come ha detto lei, che l'accordo porta, il nostro movimento con il movimento cui lei appartiene, a una rivisitazione della geografia giudiziaria. Noi le chiediamo, pertanto, di dare efficacia a questo contratto con la stessa lealtà e trasparenza che contraddistingue tutto questo Governo del cambiamento, di cui lei fa parte integrante insieme ai Ministri e insieme al Presidente del Consiglio.

le crescenti preoccupazioni che riguardano numerose famiglie e numerose imprese italiane. Dopo quattordici trimestri consecutivi di crescita, il PIL nel trimestre luglio-settembre evidenzia una prima grave stagnazione. Se inseriamo il tutto in un quadro macroeconomico che tutti gli osservatori e le autorità indipendenti, anche durante le nostre audizioni, hanno evidenziato come preoccupante per effetto di un rallentamento di un ciclo espansivo dell'economia globale, risulta evidente a tutti che non è consentito e non è sufficiente, è inadeguato per il Governo italiano limitarsi a una opposizione al passato, perché a un Governo è richiesto di garantire un presente e un futuro a questo Paese. Avete scelto di abbandonare il sentiero difficile che avevamo perseguito negli ultimi anni, che coniugava il sostegno alla crescita con il consolidamento e la credibilità dei conti pubblici. Ministro, lei sa molto bene, quale economista e uomo accademico, che la credibilità nella gestione dei conti pubblici è necessaria in tutta la pubblica amministrazione, ma diventa ancora più indispensabile per un Paese che detiene il secondo debito pubblico più alto d'Europa dopo la Grecia; un debito che va governato e, nel rapporto *deficit*-PIL, ridotto, esattamente come abbiamo cercato di fare nella legislatura precedente. Le vostre politiche, invece, hanno prodotto fin qui un isolamento insostenibile, ingiusto, fuori dalla nostra cultura dell'Italia nella dimensione europea; un'iniziativa francamente deludente, anche perché si è mostrata priva di radici fondamentali e degli anticorpi necessari. Era evidente a tutti che perfino i nazionalisti e i sovranisti non possono accedere a un'idea nuova di ristrutturazione e di rivisitazione della dimensione europea, perché i sovranisti e i nazionalisti sono orientati a costruire confini, a realizzare muri piuttosto che a costruire nuove relazioni. Con la legge di bilancio avete utilizzato la flessibilità richiesta correttamente alla Commissione europea su un terreno inadeguato; avete cioè incrementato la spesa strutturale riducendo lo spazio per gli investimenti. Avete attuato politiche assistenzialiste elettorali a scapito dei necessari investimenti nell'istruzione, nell'università, nella salute, nella ricerca, nell'innovazione e nel lavoro. Avete anteposto gli equilibri del contratto di Governo alle esigenze e alle aspettative degli italiani. Ma com'è possibile rilanciare gli investimenti, Ministro, in un quadro così negativo, con la volatilità dei titoli di Stato e l'impossibilità di collocare quantitativamente il debito, con l'aggravio dei costi degli interessi dei mutui sulle famiglie e sulle imprese, con un accesso al credito che diverrà via via più difficile? Insomma, le chiediamo quali sono le iniziative che intende adottare nella dimensione europea per ricostruire una relazione corretta con l'Europa e quali per tutelare i consumatori e le famiglie italiane. *(Applausi

nel corso dei miei precedenti interventi in Parlamento ho avuto la possibilità di osservare come i fondamentali economici dell'Italia non giustifichino i livelli attuali dello *spread*. In questo momento non credo sia necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio, ma sottolineo che il nostro sistema prevede diversi strumenti che in passato hanno già dimostrato la loro efficacia in tal senso. Ritengo che sia nell'interesse del Paese e dell'Unione europea sdrammatizzare i toni del dibattito interno ed esterno per garantire la prosecuzione del dialogo instaurato, che deve concentrarsi sugli elementi fattuali della proposta di bilancio e sugli strumenti di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui già disponiamo. Siamo convinti che l'impianto della manovra assicuri il totale controllo dei nostri conti pubblici, nei limiti della moderata politica espansiva resa necessaria dal rallentamento dell'economia europea e italiana che si intende contrastare. Crediamo, inoltre, che la strategia delineata garantisca in ogni caso anche l'obiettivo della riduzione del rapporto debito-PIL, più volte ribadito dal Governo. Ricordo che, al momento, il disegno delle misure principali della manovra è ancora in via di definizione, al fine di garantire alle stesse la massima efficacia in termini di occupazione e sviluppo. Il dialogo con le autorità europee non verte sulle priorità strategiche definite nel bilancio, che sono prerogative nazionali. Le ragioni di fondo dell'azione che il Governo sta perseguendo sono state più volte evidenziate anche in sede europea e sono ulteriormente rafforzate dal confermato rallentamento dell'economia. Con questa manovra, il Governo sta cercando di contrastare il rischio di una terza recessione dall'inizio della crisi, che potrebbe avere effetti devastanti su un tessuto sociale e produttivo già messo a dura prova da quanto accaduto finora. È nostra intenzione ribadire, nell'ambito del dialogo con l'Unione europea, che i rischi prospettati non sono limitati soltanto al nostro contesto, ma possono riguardare anche gli altri Paesi dell'Unione. Per questa ragione, sarebbe quantomeno auspicabile un riconoscimento da parte delle autorità europee della necessità di affrontare questi rischi in modo congiunto e senza pregiudizi. In tale direzione prosegue il dialogo con la Commissione, con l'obiettivo di arrivare a una soluzione condivisibile. Signor Presidente, noi abbiamo apprezzato la disponibilità del Ministro, ma le sue parole non ci hanno convinto. Il Governo ha presentato una manovra che è stata bocciata da tutti, non solo dall'Unione europea; ed è stata bocciata dai risparmiatori, che iniziano a tenersi alla larga dalle aste dei titoli di Stato. I due Vice *Premier*, in particolare il vice *premier* Salvini, hanno usato parole ironiche di fronte a quanto accaduto ieri alla Commissione europea, tirando in ballo persino Babbo Natale. Lasciate perdere: non è il momento dell'ironia, non si scherza con i risparmi, con il lavoro e con il futuro di questo Paese. *(Applausi dai prima delle elezioni, è salito a 240 all'insediamento del Governo e da due mesi è attestato intorno a 300. Non è un tema per gli speculatori finanziari: impatta sulle famiglie e sulle imprese italiane. più interessi di debito pubblico, più interessi per le famiglie e le imprese, più problemi per le banche italiane. È una vera e propria stretta monetaria, che rischia di vanificare il contenuto espansivo della manovra. Così non reggiamo. Il tema non è soltanto un dialogo, che non è mai partito, con la Commissione europea: il tema è cambiare radicalmente marcia, innanzitutto dal punto di vista del metodo, aprendo un negoziato vero con la Commissione europea, e poi del merito, cambiando l'impianto della manovra, rendendola realmente sostenibile in un'ottica di medio e lungo periodo e soprattutto efficace per rilanciare la crescita del nostro Paese.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, l'entrata in vigore tra poche settimane, dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati sta suscitando in questi giorni e nelle ultime ore forti polemiche

Imporre ora l'obbligo della fatturazione elettronica tra privati sicuramente non è un approccio costruttivo del Governo con il Paese reale, con il Paese che protesta. In questo momento l'obbligo viene visto, più che altro, come un intervento vessatorio da parte del Governo nei confronti di chi produce tutti i giorni. L'adeguamento tecnologico, quindi, viene considerato non come una semplificazione, ma come una minaccia. Noi non dobbiamo permettere tutto ciò, Ministro, e il Governo deve intervenire in questa situazione.

Anche l'entità del gettito che è stata prevista nel bilancio è stata dichiarata aleatoria da molti esponenti del Governo. Si sono iscritti in bilancio 1,9 miliardi di euro, ma sono somme assolutamente aleatorie, così come sono state definite.

più semplici da poter inserire nella fattura. Ultima, ma non per importanza, è la questione delle sanzioni, perché i nostri imprenditori sono già vessati e, se voi prevedete delle sanzioni altissime per chi sbaglia pure una virgola nella fattura,

con il documento in esame i senatori interroganti segnalano alcune criticità in merito all'introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. In merito alla richiesta di disporre termini differenziati per l'introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica in ragione delle dimensioni dell'impresa, si osserva che tale soluzione introdurrebbe elementi di notevole complessità per gli operatori nella gestione quotidiana delle fatture, con la necessità di individuare di volta in volta se il soggetto emittente, ovvero quello ricevente, rientri nelle categorie per le quali decorre l'obbligo. avviene in quanto la fatturazione elettronica è un processo simmetrico che vincola non solo il soggetto emittente, ma anche quello ricevente, a gestire come elettronica la fattura ai fini della detraibilità dell'IVA. Il quadro normativo attuale esenta dall'obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che aderiscono al regime forfettario dei minimi o le imprese agricole di piccole dimensioni. Detto regime sarà esteso, ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge di bilancio, ai contribuenti che hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi ragguagliati ad anno non superiori a euro 65.000 Con riferimento ai rilievi avanzati dal Garante della *privacy*, si fa presente che è stato attivato un tavolo tecnico congiunto tra l'Agenzia delle entrate e l'Autorità, finalizzato a individuare le soluzioni più idonee atte a superare quanto rilevato. Per quanto riguarda la disapplicazione o la riduzione delle sanzioni in caso di ritardi nell'emissione delle fatture elettroniche, è utile notare che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge fiscale collegato alla manovra di bilancio in corso di conversione, i soggetti che liquidano l'IVA su base trimestrale in relazione alle operazioni effettuate nel secondo semestre 2019 hanno la possibilità di emettere fattura elettronica entro il 20 agosto, senza applicazione di sanzioni, o entro il 16 novembre con la riduzione delle sanzioni dell'80 per intervenire in replica il senatore Damiani, perché non devono essere questi ultimi a semplificare la vita del direttore dell'Agenzia delle entrate *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*, ma dev'essere lo Stato a semplificare la vita di tutti noi cittadini. Imporre l'obbligo della fatturazione elettronica è oggi un cappio al collo ai nostri imprenditori lo può verificare direttamente dalla fattura elettronica della pubblica amministrazione, che usa in maniera distorta il rifiuto del pagamento. Ecco perché i nostri imprenditori non vengono pagati anche dalle pubbliche amministrazioni. Questi sono i problemi da risolvere del nostro Paese, signor Ministro. Volete rappresentare il Governo del cambiamento? Siatelo allora fino in fondo e abbiate il coraggio oggi di cambiare le prospettive, di ascoltare la gente, di prestare l'orecchio ai problemi reali del Paese. In siffatto modo, e oggi con questa riforma che metterà in assoluta difficoltà i nostri imprenditori, state mettendo

Lo *spread* è considerato, infatti, un indicatore della capacità di un Paese di restituire i prestiti. Il nostro debito pubblico, costituito in gran parte dai titoli emessi (Bot, Btp, eccetera), è pienamente sostenibile e credibile, nonostante i recenti e a parere degli interroganti immotivati *downgrade* di due agenzie di *rating*. Quelle stesse agenzie che, fino al giorno prima del fallimento della Lehman Brothers, valutavano con la tripla A le obbligazioni emesse da quest'ultima; molti cittadini e molte famiglie sono preoccupate per il costo dei loro mutui già in essere o di quelli che stanno contraendo; contraendo; i mutui per l'acquisto della prima casa costituiscono una parte importante del totale dei mutui erogati alle famiglie. Il montante mutui attuale ha raggiunto nel secondo trimestre 2018 il *record* storico, con un livello superiore a 318 miliardi di euro. Una famiglia italiana su due acquista l'immobile tramite mutuo bancario (e ogni anno ne vengono vendute circa 500.000); alla luce di quanto illustrato, le notizie che giungono alle famiglie dai *media* rischiano di essere fuorvianti, innescando il timore di vedersi aumentare da un mese all'altro la rata; ovviamente, chi abbia contratto un mutuo a tasso fisso ha la rata bloccata per sempre, indipendentemente da ciò che accade sui mercati finanziari; la preoccupazione maggiore colpisce le famiglie con mutui a tasso variabile: il loro timore è che possa esistere una correlazione (diretta o indiretta) tra tassi Euribor (indice collegato al tasso del mutuo variabile) e *spread* tra Btp A tal fine, le chiediamo, signor Ministro, di sapere in quale misura, in uno scenario a breve e medio termine, lo *spread* BTP-*bund* potrebbe permanere ai livelli attuali; in quale misura tali livelli di *spread* possono condizionare, seppur indirettamente, il tasso Euribor e, quindi, le rate dei mutui a tasso variabile esistenti e i mutui di nuova erogazione; in quale entità, infine, l'eventuale maggior costo della raccolta bancaria potrà trasmettersi ai nuovi mutuatari.

non solo alle scelte di politica economica, ma anche all'evoluzione del quadro economico e finanziario globale. Entrando nel merito dei quesiti rivolti dagli interroganti, per quanto riguarda l'impatto dello *spread* sui mutui ipotecari, si evidenzia che l'allargamento di tale differenziale, registrato a partire da maggio, non impatta sulle operazioni già in essere. Essi sono infatti a tasso fisso, oppure indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, che è un tasso europeo e non specifico dell'Italia. Semmai vi fosse una correlazione fra *spread* del BTP ed Euribor, essa sarebbe indiretta. Il peggioramento del differenziale sui titoli sovrani italiani può influenzare il rischio di credito sui prestiti interbancari e pertanto influenzare al rialzo anche il tasso Euribor. D'altro canto, le preoccupazioni circa la situazione italiana potrebbero far rivedere al ribasso le aspettative sui tassi di *policy* della BCE; il che, a parità di condizioni, implicherebbe un Euribor più basso. Gli andamenti registrati da maggio a oggi mostrano che l'Euribor a sei mesi è aumentato di un solo punto base (centesimo di punto percentuale), da -0,27 per cento per cento, mentre il differenziale di rendimento sui titoli di Stato italiani e tedeschi a dieci anni (lo *spread*) è aumentato di più di 180 punti base, da circa 1,3 a 3,13 punti percentuali. Per quanto riguarda, inoltre, i prestiti di nuova erogazione, gli andamenti recenti potrebbero influenzare il margine che le banche applicano sul tasso Euribor a sei mesi (mutui a tasso variabile) e il livello dei tassi a lungo termine, nel caso dei mutui a tasso fisso. I dati della Banca d'Italia, disponibili fino a settembre, indicano che, sino ad allora, lo *spread* non ha influenzato in modo avverso il livello dei tassi sui mutui. A settembre il tasso medio sulle nuove operazioni, con periodo di determinazione del tasso fino a un anno, era infatti pari all'1,51 per cento, in discesa dall'1,55 per cento di agosto e marginalmente più basso che in aprile (1,52 per cento), l'ultimo mese prima delle tensioni sul mercato dei titoli di Stato. Anche per quanto riguarda i mutui a tasso fisso, i dati Banca d'Italia mostrano che a settembre il tasso medio sulle nuove operazioni con periodo di determinazione del tasso superiore a un anno era pari all'1,93 per cento, contro il 2,0 per cento di aprile. I tassi fissi offerti alla clientela sono stati probabilmente influenzati dall'aumento del rendimento sui BTP a lunga scadenza. Tuttavia, le banche hanno traslato in modo incompleto tale aumento, riducendo i loro margini. Inoltre, la scadenza prescelta per i mutui potrebbe essere variata in qualche misura. Ciò premesso, va tuttavia segnalato che i dati di fonte ABI per il mese di ottobre indicano un aumento del tasso medio sui mutui di nuova erogazione, che l'ABI quantifica in sette punti base, all'1,87

della eventuale persistenza dell'attuale livello di *spread*, si evidenzia che, se l'aumento dello *spread* persistesse nel tempo, la traslazione sui tassi praticati dalle banche per i mutui ipotecari potrebbe risultare più significativa, come sembrano indicare i predetti dati ABI di ottobre. C'è contestualmente da notare che la principale ragione della resilienza sin qui mostrata dal sistema bancario è che la crescita dei depositi bancari è continuata fino a tutto settembre (e anche ottobre, secondo l'ABI), per cui le banche dispongono della liquidità necessaria. Inoltre, è bene ricordare che le banche sono meglio capitalizzate che in passato e hanno notevolmente ridotto il loro *funding gap* (differenza fra *stock* di prestiti erogati e raccolta tramite depositi e strumenti assimilati).

il nostro è un grande Paese, checché ne dicano altri: siamo la terza economia europea, la seconda manifattura in Europa e tra i sette Paesi più industrializzati nel mondo e, quindi, abbiamo tutte le possibilità per continuare a produrre ricchezza, assicurare benessere ai cittadini e tornare a essere *leader* economici e politici in Europa e nel mondo. *(Applausi

un immane sacrificio di vite umane. Le vittime furono circa 22.000 su una popolazione residente di circa 65.000 abitanti, quindi quasi un terzo. avvenne perché Foggia era un fondamentale snodo ferroviario (uno dei più importanti in Italia), nonché sede di piste di volo e aeroporti militari importantissimi. Appare, quindi, oggi paradossale che Foggia sia stata prima privata di un aeroporto funzionante e che poi, a poco a poco, sia diminuita la sua centralità nel traffico ferroviario, essendo diminuiti i treni che vi transitano e vi si fermano.

in Italia per estensione, la quale presenta un *deficit* enorme dal punto di vista infrastrutturale e del trasporto pubblico sia su ferro che su gomma. Per questo motivo chiedo a Trenitalia, anche a nome degli altri parlamentari del MoVimento 5 Stelle della provincia di Foggia, di rivedere questa decisione e di prevedere la fermata nella stazione di Foggia di questi e di altri treni che transitano nella città, essendo del tutto assurdo e antieconomico accettare l'idea che infrastrutture e mezzi pagati con le tasse di tutti i cittadini italiani siano posti al servizio solo di alcuni e non di altri. Non è accettabile che alcuni treni passino in un'importante capoluogo di Provincia e non vi si fermino. I cittadini di Foggia hanno espresso nelle ultime ore il loro forte disappunto e attendono risposte immediate e positive da Trenitalia. *(Applausi

Signor Presidente, signori senatori, debbo con estremo rammarico e dolore rendervi edotti dell'ennesimo femminicidio consumatosi a Sala Consilina, in provincia di Salerno, circa quindici giorni fa. Una giovanissima donna e mamma affettuosa di tre bambini in tenerissima età è rimasta vittima di un efferato delitto. L'autore non ha esitato a rovesciarle addosso un'intera tanica di benzina e a darle fuoco. Il raccapricciante delitto ha scosso l'intera comunità di Sala Consilina e ancora oggi in paese aleggiano un velo di sgomento, stupore e tristezza uniti a un forte senso di vicinanza e di cordoglio nei confronti dei familiari. È stato un atto criminoso e brutale, commesso in totale violazione dei diritti umani. Ci si sforza, da buoni cristiani, di trovare una giustificazione, ma l'orrore è tanto grande da non poterlo consentire. Ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa da un marito, un fidanzato, da un compagno o un ex compagno di vita. Le cause sono generate da un forte senso di insicurezza, da un desiderio di dominio psicologico sulla donna schiavizzata, da comportamenti violenti e prevaricatori dal non volersi assuefare alla condizione di un eventuale abbandono; mentre, dall'altro canto, c'è la donna smarrita, sottomessa, incapace di trovare il coraggio di denunciare e porre fine all'immeritato supplizio. Questo problema è diventato universale e riguarda tutti, e non solo coloro che a vario titolo sono stati vittime dirette o indirette di tali efferatezze. È stata, non a caso, istituita una giornata mondiale contro la violenza sulle donne, affinché il sacrificio di tante vittime innocenti non risulti vano. Adesso bisogna ragionare in termini di vera e propria emergenza sociale e il problema deve essere affrontato alla radice, coinvolgendo tutti, privati cittadini, istituzioni e soprattutto la scuola, la quale deve svolgere un ruolo primario e imprescindibile al fine di inculcare nella mente dei giovani il rispetto per il prossimo, la sacralità della vita e la libera e pacifica convivenza tra tutti i consociati. Purtroppo, troppo spesso l'amore e la dedizione verso un marito o un compagno vengono ripagati con la perdita della vita. Finora qualcosa si è mosso a livello istituzionale, signor Presidente e signori senatori, ma non basta, visti gli ultimi efferati eventi. Oggi, ripaghiamo con violenza e orrore colei che cristianamente ha fatto suo il messaggio di Cristo e in quell'amore ha creduto; ha vissuto ricevendone in cambio, come agnello sacrificale, una morte È giunto il momento di ribellarci a tutto ciò e poniamo una volta per tutte fine a questo abominio.

un fare in fretta, il più in fretta possibile da parte dei partiti di maggioranza. Mi limito a segnalare alla Presidenza che, per il rispetto che dobbiamo a questa istituzione e al rapporto tra le due Camere,